L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Senatore Battaglia, a fine seduta potrà tornare sull'argomento.

il provvedimento in titolo, d'iniziativa governativa, reca le consuete disposizioni di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore dell'Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali, con Allegati, fatto a Ginevra il 27 gennaio 2006. Quanto ai contenuti dell'Accordo, ricordo in premessa che l'Organizzazione internazionale sui legni tropicali

Il passo iniziale fu costituito dalla Conferenza di Nairobi del 1976, che stabiliva un piano d'azione per la strutturazione del commercio dei prodotti di base. I successivi negoziati hanno condotto all'Accordo del 1983 e, successivamente, all'attuale Accordo internazionale sui legni tropicali del 1994, che rimarrà valido fino all'attuazione del successivo Accordo ITTA del 2006, di cui al disegno di legge di ratifica in esame. L'Accordo ITTA 2006 si propone la realizzazione di programmi di ricerca e di sviluppo, la commercializzazione e la distribuzione del legname tropicale, la gestione forestale e il mantenimento dell'equilibrio ecologico nelle zone interessate. Per l'attuazione dell'accordo rimane in essere l'Organizzazione internazionale dei legni tropicali Organization*) che esercita le sue funzioni attraverso il Consiglio internazionale dei legni tropicali, organo direttivo costituito da tutti i Paesi membri produttori e consumatori. Al Consiglio si aggiungono il direttore esecutivo, i comitati permanenti e gli organi ausiliari. Tra i comitati permanenti, aperti a tutti gli Stati membri e gli osservatori, rientrano il comitato per le questioni economiche, le statistiche ed i mercati; il comitato per il rimboschimento e la gestione forestale; il comitato per l'industria forestale; il comitato finanziario e amministrativo. Quanto ai contenuti dell'Accordo, l'articolo 1 ne indica gli obiettivi, quali, nel rispetto di una gestione forestale sostenibile, la lotta alla povertà e all'illegalità delle pratiche di deforestazione nei Paesi produttori. elencano competenze e mansioni, precisano le funzioni relative alle cariche del presidente e del vice presidente. Gli articoli 10, 11, 12 e 13 illustrano la ripartizione dei voti tra Paesi produttori e Paesi consumatori, specificandone i criteri di assegnazione e la procedura di voto. Gli articoli 15 e 16 fanno riferimento alla cooperazione tra l'organizzazione ITTO e gli organi e le agenzie delle Nazioni Unite, nonché istituzioni internazionali e regionali, organizzazioni non governative, settore privato e società civile. Viene anche disciplinata l'ammissione di osservatori. Gli articoli 18, 19, 20 e 21 istituiscono i conti finanziari e la rispettiva metodologia di calcolo, distinti in: «conto amministrativo», «conto speciale» e «fondo per il partenariato di Bali». Segnalo che dette disposizioni costituiscono, infatti, la principale novità rispetto al previgente Accordo. In particolare, il conto amministrativo è finanziato dai contributi annui fissati per ciascun Stato membro, in conformità alle rispettive procedure costituzionali o istituzionali e comprende i costi amministrativi di base (stipendi i costi operativi essenziali (a copertura di riunioni di esperti, pubblicazioni di studi e valutazioni); il conto speciale è destinato a finanziare programmi tematici e i contributi ad esso destinati rivestono carattere volontario da parte dei Paesi membri; il fondo per il partenariato di Bali consiste in un deposito speciale destinato a sostenere e incrementare gli investimenti dei Paesi membri produttori e viene finanziato dai contributi dei Paesi membri donatori e dal 50 per cento dei proventi delle attività correlate al conto speciale. Sulla base delle determinazioni assunte in sede comunitaria, si è stabilito l'impegno della Comunità europea ad erogare il contributo finanziario obbligatorio al conto amministrativo. Pertanto, con l'entrata in vigore del nuovo accordo, gli impegni finanziari obbligatori verranno assunti direttamente dalla Comunità europea, in funzione del volume delle importazioni di legname tropicale di ciascuno Stato membro dell'Unione europea. Gli Stati membri saranno dunque esentati dal versamento di qualunque onere di spesa di natura obbligatoria. Per quanto riguarda il pagamento da parte italiana di contributi finanziari volontari da destinare al bilancio del conto speciale per interventi su specifici progetti, si tratta di un'ipotesi eventuale da finanziare con apposito disegno di legge. Dal provvedimento non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

che non presenta peraltro incompatibilità con altre leggi, ma, anzi, le sostiene ampiamente, anche nel rispetto del Trattato di Lisbona e nell'ambito dei cambiamenti climatici e della lotta alla desertificazione. Dall'attuazione del provvedimento scaturiscono quindi per l'Italia benefici sia finanziari sia commerciali sia ambientali. In termini finanziari, attraverso l'abbattimento degli attuali oneri dovuti all'Organizzazione, che verrebbero sostituiti da un unico contributo erogato a livello comunitario. In termini di tutela ambientale, il nuovo Accordo determina un miglioramento dell'opera di salvaguardia ambientale, finora garantita con l'Accordo ITTA del 1994, nel quadro di una gestione sostenibile delle esportazioni, importazioni e riesportazioni di materiali grezzi,

*(IdV)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, la deforestazione globale continua. Secondo le stime dell'OCSE, ogni anno scompare una foresta originaria delle dimensioni della Grecia. Il disegno di legge che ci apprestiamo a votare concerne un settore commerciale con un giro d'affari di miliardi di euro, che è tuttavia strettamente interconnesso alle principali emergenze ecologiche del pianeta. La produzione di legno tropicale è uno dei fattori principali della distruzione delle foreste nel mondo e meno alberi significa meno capacità di assorbimento. La concentrazione dei gas serra nell'atmosfera cresce sia per l'aumento delle emissioni sia, nel caso dell'anidride carbonica, per la sistematica distruzione di milioni di ettari di foresta: gli alberi, infatti, agiscono da veri e propri accumulatori di carbonio, e per ogni ettaro di foresta bruciato cresce quindi di un po' la quantità di anidride carbonica liberata nell'aria, e con essa l'effetto serra. Dunque, è necessaria una visione sempre più unitaria, globale se vogliamo, di problemi che riguardano alla fine tutti noi, nessuno escluso, la quale deve sfociare in politiche nazionali indirizzate verso la conservazione delle foreste tropicali e delle risorse genetiche ed al mantenimento dell'equilibrio biologico nelle regioni interessate. Noi dell'Italia dei Valori diamo un'assoluta priorità alle istanze di mantenimento dell'equilibrio ecologico e naturalistico ed agli obiettivi di protezione dell'ambiente da fenomeni di deforestazione. Allo stesso tempo il nostro Gruppo conserva il realismo dettato dalle considerazioni economiche, per cui specifiche attività produttive, che risultano preziose sotto il profilo dell'impiego di lavoratori e dal punto di vista dello sviluppo commerciale, devono comunque essere incentivate, cercando quindi un equilibrio fra rispetto di standard ambientali e *input* produttivi. L'Accordo internazionale che ci accingiamo ad accogliere nel nostro ordinamento si prefigge, tra le altre cose, di istituire un foro di consultazione tra Paesi produttori e Paesi consumatori, di favorire la cooperazione internazionale, l'elaborazione di linee politiche relative all'economia mondiale del legno e l'adozione di pratiche non discriminatorie nel commercio del legname. Signora Presidente, colleghi, alcuni punti ambigui devono purtuttavia essere menzionati. L'articolo 1, che fissa gli obiettivi dell'Accordo del 2006 e dei precedenti, parla in primo luogo di «favorire l'espansione e la diversificazione del commercio internazionale», menzionando solo in seguito la sostenibilità.

sono determinati prevalentemente dalle loro importazioni medie nette di legni tropicali. Pertanto, malgrado tutta la retorica sulla sostenibilità, il sistema è concepito per attribuire la massima influenza ai Paesi che maggiormente commerciano. Di non secondaria rilevanza, secondo noi, è il fatto che la struttura dell'Accordo abbia un'impronta fortemente governativa, poiché non attribuisce alcun ruolo esplicito ai parlamentari o alla società civile nella formulazione delle politiche. Ad ogni modo, attribuiamo importanza a questa iniziativa che rappresenta un primo passo verso una più oculata gestione del patrimonio forestale. Ugualmente, riteniamo che si debbano perseguire obiettivi ancora più ambiziosi giungendo, appena possibile, all'apertura di negoziati per la firma di una convenzione mondiale che stabilisca uno strumento giuridico vincolante per la gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, non solo quindi quelle tropicali. Qualsiasi accordo dovrebbe essere inserito in un approccio più generale, che contempli anche le foreste delle zone temperate, la domanda di prodotti derivati dal legno e la tracciabilità lungo l'intera filiera di approvvigionamento. L'approvazione da parte del Parlamento di questo disegno di legge deve essere intesa dall'Italia dei Valori come l'avallo di un Accordo tutto sommato insoddisfacente. Occorre riconoscere, infatti, che il risultato ottenuto è di gran lunga inferiore a quanto necessario per affrontare il problema della perdita delle foreste tropicali. Tuttavia, considerando l'atto come la presa di coscienza di un problema evidente, voteremo a favore nella speranza di una cooperazione internazionale sempre più profonda nel settore. *(Applausi dei

l'Italia ha ratificato, come ultimo Stato firmatario, la Convenzione per la protezione delle Alpi. Essa reca il riconoscimento, tra Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Principato di Monaco, Slovenia e Svizzera, del concetto delle Alpi come una vasta area unitaria nel centro dell'Europa che, per le sue particolari caratteristiche ambientali e culturali, richiede una capacità di pianificazione e di intervento e una protezione dell'ecosistema alpino a carattere sovranazionale. Con la Convenzione si persegue la salvaguardia a lungo termine dell'ecosistema naturale delle Alpi e lo sviluppo sostenibile dell'area alpina, oltre alla tutela degli interessi economici delle popolazioni residenti, stabilendo i princìpi cui dovrà ispirarsi la cooperazione tra i Paesi dell'arco alpino in alcuni settori prioritari, tra cui la pianificazione territoriale, la difesa del suolo, la tutela del paesaggio, l'agricoltura di montagna, la protezione della natura, le foreste montane, il turismo e il tempo libero, i trasporti, l'energia e i rifiuti. Per dare attuazione alla Convenzione delle Alpi è necessario adesso ratificare alcuni importanti Protocolli attuativi già predisposti da gruppi di lavoro insediati dai Paesi firmatari della Convenzione, come previsto dall'articolo 2 della stessa, e firmati dai Ministri dell'ambiente in un arco di tempo che va dalla III Conferenza delle Alpi tenutasi a Chambéry il 12 dicembre 1994 fino alla VI Conferenza delle Alpi, che si è riunita a Lucerna, in Svizzera, il 30-31 ottobre 2000. I Protocolli da ratificare sono i seguenti. 1. Il Protocollo sulla protezione della natura e la tutela del paesaggio, al fine di proteggere, curare e ripristinare, se necessario, lo stato naturale ed il paesaggio, in modo da assicurare l'efficienza funzionale degli ecosistemi, la conservazione degli elementi paesaggistici e delle specie animali e vegetali selvatiche insieme ai loro *habitat* naturali. Il Protocollo sull'agricoltura di montagna prevede principalmente di incentivare l'agricoltura di montagna anche sulla base delle peculiarità delle zone montane nell'ambito della pianificazione territoriale, della destinazione delle aree, del riordinamento e miglioramento fondiario. 3. Il Protocollo su pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile prevede l'elaborazione di strumenti articolati di pianificazione a livello locale, al fine di coordinare gli aspetti dello sviluppo con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente, consentendo uno sviluppo regionale che offra opportunità di lavoro alle popolazioni interessate. 4. Il Protocollo sulle foreste montane contempla la predisposizione di strutture di base per la pianificazione forestale, garantendo le funzioni protettive delle foreste 5. Il Protocollo sull'energia è teso a migliorare la compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia nell'arco alpino, anche mediate i risparmi ottenuti attraverso la razionalizzazione dell'energia stessa. 6. Il Protocollo sulla difesa del suolo prevede che i terreni meritevoli di protezione siano inclusi nelle aree protette, considerata l'indubbia rilevanza della loro buona conservazione, e che si debba dare luogo ad un uso contenuto del terreno, nonché delle risorse minerarie e delle attività estrattive. 7. Il Protocollo sul turismo persegue l'obiettivo di contribuire ad uno sviluppo sostenibile del territorio alpino attraverso un turismo rispettoso dell'ambiente; le parti sono impegnate ad adottare specifici provvedimenti e raccomandazioni che non trascurino gli interessi né della popolazione locale né dei turisti. 8. Il Protocollo sui trasporti, le cui trattative sono iniziate nel 1994, ha presentato particolare difficoltà nella predisposizione del testo, stante la delicatezza degli aspetti economici ed ambientali, concernendo una regione di passaggio, come quella alpina, che presenta le peculiarità e le esigenze di tutela a tutti ben note. Questo è stato uno degli argomenti a causa dei quali si è arrivati solo oggi all'approvazione di questi Protocolli. 9. Il Protocollo sulla composizione delle controversie è teso a colmare una lacuna della Convenzione base attraverso l'introduzione di particolari meccanismi in caso di divergenti interpretazioni delle disposizioni della Convenzione stessa o dei Protocolli successivi. Il disegno di legge governativo n. 1474, assunto come testo base e approvato dalla Commissione in sede referente, reca le disposizioni di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore dei suddetti Protocolli. Avevano il medesimo contenuto Avevano il medesimo contenuto anche gli assorbiti disegni di legge n. 22, d'iniziativa dei senatori Peterlini e altri, e n. 381, presentato dai senatori Della Seta ed altri. Dette proposte legislative differivano invece con riferimento alla clausola di quantificazione degli oneri e modalità di copertura finanziaria. Ricordo peraltro che le citate iniziative legislative riproducono i disegni di legge presentati dal Governo, di ratifica ed esecuzione di tutti i Protocolli di attuazione della Convenzione, già nelle due passate legislature. Nella XIV legislatura l'*iter* del provvedimento non si era concluso, sino alla sospensione dell'esame da parte delle Camere. Il testo era giunto alla seconda lettura da parte della Camera dei deputati privo del Protocollo sui trasporti, come ricordavo prima. Ciò fa comprendere la presentazione, nella presente legislatura, anche degli assorbiti disegni di legge n. 47, d'iniziativa dei senatori Peterlini e altri, e n. dalla senatrice Thaler Ausserhofer, di identico contenuto e recanti l'autorizzazione alla ratifica del solo Protocollo «trasporti» allegato alla Convenzione. Vorrei ora svolgere alcune brevi considerazioni di carattere personale. In primo luogo, le Alpi rappresentano per il turismo un'autentica risorsa: l'Organizzazione mondiale per il turismo informa che questa vasta area accoglie ogni anno circa il 12 per cento del turismo mondiale. Inoltre le Alpi rappresentano anche uno dei più vasti patrimoni di diversità biologica in Europa, con ben 30.000 specie animali e 13.000 specie vegetali. Già solo questi due dati spiegano bene l'importanza di addivenire finalmente, dopo troppi anni di *impasse*, alla ratifica da parte italiana dei Protocolli. In secondo luogo, la Convenzione sulla protezione delle Alpi del 1991 rappresenta uno strumento ancora vivo e tutt'altro che obsoleto (ma solo a patto che finalmente i Protocolli vedano una piena attuazione in tutti i Paesi firmatari). Lo dimostrano le intense attività del suo segretariato, che per i prossimi due anni sarà affidato alla Slovenia, e la produzione di studi importanti, come quello dell'anno scorso sui trasporti e sulla mobilità nelle regioni alpine o come quello sull'acqua, adottato lo scorso marzo dalla Conferenza dei Ministri dei Paesi aderenti a Evian, in Francia. In terzo luogo, infine, le Alpi non sono solo una grande attrazione turistica e naturalistica. Esse hanno, infatti, un enorme valore sul piano climatico, il che, detto per inciso, ha anche un significato ulteriore proprio in occasione del G8 dei Ministri dell'ambiente, ospitato a Siracusa. In tal senso si spiega perché, ancora a Evian, lo scorso 12 marzo, i Governi dei Paesi aderenti alla Convenzione abbiano adottato un Piano d'azione sul cambiamento climatico nelle Alpi, che pone una serie di obiettivi sui vari piani, a partire da quelli delle fonti energetiche rinnovabili e della preservazione della biodiversità. Questo contesto generale spiega bene perché sia urgente che, dopo i tentativi andati a vuoto per le più varie ragioni nelle scorse due legislature, il Parlamento arrivi ora ad una sollecita ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione alla Convenzione per la protezione delle Alpi. Non bisogna poi dimenticare un risvolto che è anche di carattere culturale: le Alpi rappresentano infatti una grande area che accomuna popolazioni appartenenti a Nazioni diverse grazie all'affermazione di una vera e propria cultura della montagna, che ha fatto prevalere i sentimenti dell'amicizia e della comprensione rispetto a quelli, pur presenti in un passato ancora recente, dell'incomprensione e della diffidenza reciproca. Auspico quindi l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento in esame.

che, in base a quanto evidenziato dal relatore, rivestono una grandissima importanza in campo economico, ambientale e sociale per l'arco alpino e per tutta l'Italia.

di presiedere importanti gruppi di lavoro e di vedere il ruolo di segretario generale affidato a un connazionale, il dottor Marco Onida, peraltro di lunga esperienza comunitaria.

prendo brevemente la parola per esprimere, a nome del Gruppo dell'Italia dei Valori, pochi semplici concetti e qualche auspicio in favore dell'atto di cui discutiamo. Come sappiamo, l'Italia ha ratificato nel 1999 la Convenzione per la protezione delle Alpi, che era stata firmata otto anni prima a Salisburgo. Tale Convenzione reca il riconoscimento - tra Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Principato di Monaco, Slovenia e Svizzera - dell'arco alpino come una vasta area unitaria che, per le sue particolari caratteristiche ambientali e culturali, richiede interventi concertati a livello sovranazionale. Detta Convenzione tende alla salvaguardia dell'ecosistema delle Alpi nell'ambito e in applicazione di princìpi, come lo sviluppo sostenibile, oltre che alla tutela degli interessi economici delle popolazioni residenti. individua ben 12 settori sui quali tale cooperazione tra gli Stati dovrà enuclearsi. La pianificazione del territorio, la difesa del suolo e del paesaggio, il turismo, lo studio dei trasporti, l'uso dell'energia e dei rifiuti sono, almeno per quello che ci possibile apprendere da questo testo, i punti salienti, ovvero i Protocolli su cui gli organi previsti dalla suddetta Convenzione dovranno confrontarsi e porre in essere atti concreti, con gli aiuti dei Ministeri dell'ambiente di ogni singolo Paese, al fine di tutelare lo spettacolare ecosistema rappresentato dalla catena alpina. La Convenzione prevede inoltre l'istituzione della Conferenza delle parti contraenti e, al suo interno, un Comitato permanente che, di fatto, sarà l'organo esecutivo ristretto. Spero che la previsione della convocazione di tale Conferenza solo una volta ogni due anni non risulti insufficiente a sortire gli effetti sperati o addirittura causa di nocumenti a chi in quella zona stupenda del continente vive, lavora e si adopera da sempre per il corretto sfruttamento del territorio. Concludo, signora Presidente, chiedendo al Governo di adoperarsi affinché i rappresentanti italiani che siederanno negli organi su richiamati perseguano questi obiettivi ambiziosi. tutela del territorio e del mare e a quello degli affari esteri di produrre tutto il loro sforzo affinché i soliti ritardi burocratici non vadano ad intaccare la funzionalità di una Conferenza e dei suoi organi, che già in partenza

tra tutti i Paesi che hanno firmato e ratificato la Convenzione, è quello che vanta la più ampia superficie del territorio alpino considerato. Questo provvedimento colma davvero una lacuna

in un territorio complesso, che non è possibile spezzettare tra i vari Paesi che lo custodiscono, bisogna inevitabilmente e necessariamente porsi in un'ottica di governo sovranazionale. Questa è la scommessa che ormai molti anni fa

del territorio alpino, anche ambiti che hanno molto a che fare con lo sviluppo sostenibile. Cito soltanto il caso dei trasporti: il Protocollo sui trasporti è stato uno di quelli che più faticosamente hanno camminato in questi anni. Molto spesso ragioniamo e discutiamo di grandi infrastrutture di trasporto (penso al corridoio 5, Lisbona-Kiev), che

consentono di gestire e realizzare in maniera più uniforme e, credo, anche più efficace. L'ambiente, tra tutti temi in cui si esercita la politica, è forse quello che richiede maggiormente

il provvedimento in titolo, d'iniziativa governativa e già approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura senza modificazioni, reca le consuete disposizioni di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore dello Scambio di Note intercorso tra il Governo italiano e il Consiglio federale elvetico sul reciproco confine. in questione risale al mese di maggio 2008 e ha per oggetto il confine tra le due Nazioni, che si trova lungo l'arco alpino che separa l'Italia e la Svizzera, dalla Valle D'Aosta fino al Trentino. Si tratta di zone di alta montagna di proprietà demaniale e, quindi, non si produrranno conseguenze di alcun tipo per gli abitanti delle zone di confine come singoli, che invece potranno fruire ulteriormente dei buoni rapporti bilaterali tra i due Stati. La linea di confine tra l'Italia e la Svizzera è stata individuata mediante rilevazioni e misurazioni che si sono concluse nel 1941, anno in cui è stata sottoscritta a Berna un'apposita Convenzione e il relativo regolamento. In tal modo sono stati disciplinati nel tempo i lavori di manutenzione ai termini del confine. La manutenzione ha consentito negli anni di individuare visivamente i riferimenti morfologici del confine italo-svizzero, per esempio, i cippi collocati lungo la linea di demarcazione. fattori climatici e ambientali, come anche la riduzione della superficie dei ghiacciai e dei nevai perenni, hanno compromesso negli anni l'evidenza fisica della linea di confine eliminando i punti di riferimento morfologici stabiliti con la citata Convenzione del 1941. Si è quindi posta l'esigenza per la Commissione per la manutenzione del confine italo-svizzero, riunitasi ad Aosta il 10 e 11 novembre 2004, di sostituire ai riferimenti originari una diversa modalità di individuazione del confine tra i due Stati, la quale fa riferimento ad una nuova nozione di frontiera, non più rigidamente fissa, bensì in dipendenza dei graduali cambiamenti provocati dall'erosione e dalla contrazione dei ghiacciai, fino al caso limite della loro scomparsa. la linea di demarcazione diviene mobile e coincide con la cresta del ghiacciaio o con la linea di cresta del terreno roccioso emergente, laddove il ghiacciaio stesso sia scomparso. Ciò anche in previsione di ulteriori mutamenti di temperatura. Per linea displuviale si intende, invece, la linea sulla quale si separano sul terreno le acque del deflusso, senza considerare le infiltrazioni d'acqua negli strati inferiori del terreno. Ove si verificassero, invece, non erosioni o cambiamenti graduali, ma modificazioni repentine o superficiali della linea displuviale o della linea di cresta, non si produrrà automaticamente alcun cambiamento del tracciato del confine e in tal caso Italia e Svizzera potranno eventualmente prevedere uno scambio di superfici equivalenti. La linea di frontiera così definita sarà individuata tramite appositi rilievi e resterà così fissata fino ai rilievi successivi. Sulla base delle considerazioni che precedono, si auspica l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento in esame.

con la ratifica da parte del Parlamento italiano. Con la Francia le trattative per la conclusione di un analogo Scambio di Note sono state già avviate, mentre con la Slovenia il problema non sussiste dato che non ci sono ghiacciai. Quindi, il Governo sollecita la rapida ratifica da parte del Parlamento di questo provvedimento, anche in considerazione della valenza politica dei nostri rapporti bilaterali con la Svizzera

Signora Presidente, colleghi, signora Sottosegretario, l'Italia dei Valori voterà a favore

è particolarmente importante perché non solo i cambiamenti climatici ci sono, eccome, rispetto al passato, ma essi influiscono pesantemente addirittura sul concetto di sovranità e sul suo esercizio da parte di uno Stato. Come sappiamo, le zone di confine riguardano terreni demaniali il cui accesso è difficile se non, talvolta, impossibile. Ricordo di aver studiato, molti anni addietro, che nelle zone di montagna i confini si calcolavano con specifiche modalità che necessariamente dovevano dipendere da fattori quali l'altezza e la posizione della cresta dei ghiacciai o delle linee di cresta del terreno roccioso emergente. Ho inoltre appreso, sempre leggendo questo di disegno di legge di ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra Italia e Svizzera, che i suddetti cambiamenti climatici impediscono oggi di individuare visivamente i riferimenti morfologici del confine italo-svizzero stabiliti dalla Convenzione di Berna del 1941 (come è detto testualmente nella relazione "cippi collocati lungo la linea di demarcazione"). Concludo, quindi, signora Presidente, con l'auspicio che gli Stati, Stati, tutti, a prescindere dal problema di confine, si adoperino al fine di contenere i cambiamenti climatici e di preservare la natura, così come abbiamo la fortuna di poterne usufruire oggi. Anche se in questo caso agito con meno ritardo rispetto ad altri atti di ratifica, mi auguro che trattati bilaterali come questo, o addirittura semplici Scambi di Note, possano trovare più celere attuazione al fine di poter produrre quanto prima gli effetti sperati. L'Italia dei Valori, quindi, voterà a favore. Presidente, in Commissione abbiamo lungamente Grazie

Signor Presidente, il provvedimento in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, si compone di tre articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo che modifica che modifica la Convenzione relativa all'Organizzazione idrografica internazionale, fatto a Monaco Principato il 4 luglio 2005. Viene poi disposta l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. L'Organizzazione idrografica internazionale (IHO), con sede nel Principato di Monaco, è un organismo intergovernativo di carattere tecnico e consultivo che è succeduto all'Ufficio idrografico internazionale, che era sorto nel 1921. Attualmente aderiscono all'Organizzazione circa 80 Stati membri, tra cui l'Italia, che ha ratificato la Convenzione istitutiva con legge 15 novembre 1973, I principali scopi perseguiti dall'Organizzazione, elencati all'articolo II della Convenzione, sono: il coordinamento delle attività degli uffici idrografici internazionali; la maggiore uniformità possibile nelle carte e nei documenti nautici; l'adozione di metodi sicuri ed efficienti per l'esecuzione e l'utilizzazione dei rilevamenti idrografici; lo sviluppo delle scienze nel campo dell'idrografia e delle tecniche impiegate per i rilevamenti oceanografici. La struttura interna dell'Organizzazione include l'Ufficio idrografico internazionale (IHB), amministrato da un Comitato direttivo e la Conferenza, organo assembleare che riunisce i rappresentanti dei Governi membri. All'interno dell'Organizzazione l'Italia è rappresentata dall'Istituto idrografico di Stato, ente della Marina militare, che ha sede a Genova. Il Protocollo in esame, composto di 20 articoli ed approvato nel corso della Conferenza straordinaria di Montecarlo dell'11-15 aprile 2005, apporta profonde modifiche alla Convenzione ed è diretto a cambiare la struttura dell'IHO rendendola più simile a quella di altre organizzazioni internazionali quali l'IMO (*International Marittime Organization*) e l'IOC (*Intergovernmental Oceanographic Commission*). Non entro nel merito dell'articolato, rinviando alla relazione scritta che consegnerò alla Presidenza. Per l'importanza di questo organismo e trattandosi soltanto di un adeguamento e di un rinnovamento della sua struttura organizzativa, chiedo e auspico l'approvazione da parte dell'Assemblea. il Protocollo di modifica della Convenzione, pur configurandosi come una rivisitazione profonda, mantiene una struttura giuridica simile a quanto già in essere e lo stesso personale; di conseguenza, non comporta alcun aggravio di oneri finanziari. Dal provvedimento continueranno a derivare benefìci per l'Italia in termini di sicurezza della navigazione e tutela dell'ambiente marino, in conseguenza della condivisione, in ambito internazionale, delle più moderne tecniche scientifiche di rilevamento e dei relativi dati idrografici.

della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990,

Grazie La citata Convenzione si applica alle imposte sui redditi quando gli utili di una impresa rischiano di ricadere contemporaneamente nella imposizione fiscale di due Stati contraenti. Ciò può avvenire poiché, ove la sede di un'impresa sia situata in un Paese diverso da quello della casa madre, ricade nella disciplina fiscale dello Stato in cui è situata. Tralascio le ipotesi. Il 25 maggio 1999 è stato concluso dagli Stati allora componenti dell'Unione il Protocollo di modifica della Convenzione del 1990, per cui il termine di durata della stessa, previsto originariamente in cinque anni dall'entrata in vigore, è stato automaticamente prorogato per periodi quinquennali, salvo il caso di obiezioni di una delle si è verificato l'allargamento dell'Unione europea ad otto Paesi dell'Europa centro-orientale, oltre a Malta e Cipro, e ciò ha comportato per i dieci nuovi membri l'impegno a divenire parti della citata Convenzione del 1990. 1990. La Convenzione del 2004, oggetto del disegno di legge di ratifica in esame, ha tale precipua finalità. Essa è già entrata progressivamente in vigore nei rapporti bilaterali tra gli Stati membri che hanno depositato i pertinenti strumenti di adesione, senza necessità del raggiungimento di un numero minimo di ratifiche. di sette articoli, il primo dei quali prevede l'adesione dei dieci Stati entrati a far parte dell'Unione europea nel 2004 alla Convenzione del 1990. L'articolo 2, comma 1, integra l'elenco delle imposte dei Paesi aderenti alle quali si applica la Convenzione del 1990, includendovi alcune imposte dei dieci nuovi Paesi, ma anche - come è il caso dell'Italia con l'IRES e l'IRAP - categorie di imposte nel frattempo intervenute anche con riferimento a Stati già membri dell'Unione.

Stato membro dell'Unione a non aver ancora concluso l'*iter* di ratifica. L'impegno politico deriva dal codice di condotta per l'effettiva attuazione della Convenzione sull'arbitrato adottato nel 2006 dal Consiglio dell'Unione europea, con il quale gli Stati membri si sono impegnati a firmare e ratificare la Convenzione in questione il più presto possibile e, in ogni caso, entro due anni dall'adesione all'Unione di nuovi Paesi. La Convenzione costituisce un utile strumento per il superamento, in ambito comunitario, dei problemi in materia di doppia imposizione. La sua estensione ai nuovi Paesi membri contribuisce sicuramente al miglioramento del quadro di riferimento per gli operatori economici.

Esso fa solo una cosa: funziona. Così, in questo nostro mondo, ormai corrosi dal nichilismo, i concetti di individuo, di identità, di libertà, di senso, ma anche quelli di natura, di etica, di politica, di religione, di storia, di cui si è nutrita tutta l'età pre-tecnologica, finiscono sullo sfondo della società. Chi però paga di più la sostanziale assenza di futuro sono i giovani, che rischiano di vivere parcheggiati in una terra di nessuno, dove la famiglia e la scuola non dialogano più, dove il tempo è vuoto e dove è sempre più difficile creare un «noi» motivazionale. La società in cui viviamo, di cui la scuola è una delle componenti fondamentali, è coinvolta in una crisi grave, che oltre che economica e politica è anche sociale, ma è soprattutto culturale, innescata in parte dai veloci meccanismi della globalizzazione, che sembrano però aver pesato sul sistema Italia più che sugli altri Paesi europei. Se prendiamo in considerazione i risultati delle tre indagini PISA-OCSE, è evidente sia il ritardo nei vari settori disciplinari degli studenti italiani rispetto a quelli europei, europei, sia una crisi generalizzata della scuola italiana nel suo complesso, che si riflette in un evidente arretramento culturale della società, in uno scadimento generale dei valori, dei comportamenti, del rispetto delle regole, del senso di appartenenza ad una comunità. Eppure, l'Agenda di Lisbona ci ha invitati a costruire "la società più dinamica e competitiva del mondo" della scienza e della conoscenza; ma quanto siamo disposti ad investire per raggiungere questo ambizioso obiettivo? Perché i nostri giovani siano in grado di affrontare le nuove sfide che impone una società sempre più complessa? Se è vero com'è vero che le sfide globali possono essere affrontate, e vinte, soltanto a livello di continenti e non più come Paesi, ciò comporta per il nostro Governo, come per gli altri Governi europei, l'obbligo di assumere la cultura e la formazione dei giovani come priorità su cui investire con convinzione per ridurre il nostro *gap* culturale e tecnologico. Occorre che il Governo intensifichi lo sforzo economico per una scuola di qualità sotto il profilo culturale, formativo ed educativo. Il nostro tempo, signora Sottosegretario, richiede cultura, competenza, sapere e saper fare, chiavi di accesso che possono aprire le porte del mondo ai nostri figli, come la conoscenza delle lingue, il sapere scientifico tecnologico e matematico, una robusta cultura generale, la padronanza critica dei mezzi di comunicazione informatica e telematica. La scuola è infatti chiamata ad operare in un contesto ambientale caratterizzato sempre più dal rapido sviluppo tecnologico, dal dilagare di una cultura "mordi e fuggi", dall'immagine del "bla bla bla", dei moderni mezzi di comunicazione con cui non sa e non può competere, se non riformandosi radicalmente negli ordinamenti, nei metodi, nei programmi e soprattutto nel suo mezzo fondamentale di espressione culturale, che sono i libri di testo, con nuovi essenziali contributi disciplinari al passo con la modernità, con le scoperte scientifiche e in grado di supportare gli studenti nelle attività di ricerca e di elaborazione, di dare consapevolezza ed esperienza, conoscenza riflessa e soprattutto capacità critica. Sappiamo, però, che c'è un blocco fondamentale per quanto riguarda le adozioni dei libri di testo di circa sei anni e ci sono cinque anni di blocco anche per riformare i contenuti degli stessi libri di testo in variazione. Tutto questo cozza anche con una pseudoriforma che deve decollare entro il 2010, soprattutto degli istituti tecnici, che a variazione del *curriculum* non vedranno variati i testi che consentiranno di procedere nel *curriculum* stesso. Chiedo quindi al Governo di intervenire assolutamente soprattutto su questo percorso. Solo la lettura, a nostro avviso, l'impegno culturale, l'accostamento critico a testi di diversa impostazione, la capacità di usare nuove tecnologie come mezzo e non come fine, per evitare il rischio di una dipendenza brutale, possono far crescere i nostri giovani e l'intera società, renderla più consapevole delle scelte equilibrate, dialogante verso culture e civiltà diverse e tradizioni altre. Sostengo da tempo, Presidente, che l'ignoranza è la più grande delle povertà e che la povertà è la madre di tutti i conflitti e di tutte le guerre, ed è per questo che dobbiamo combattere l'ignoranza per combattere la povertà. La globalizzazione ci ha portati a preferire la comunicazione telematica, la lettura di pagine *web*, limitate ad informazioni essenziali, piuttosto che quella più impegnativa dei libri. Ciò comporta vantaggi, ma forse anche forti rischi nei confronti di una superficialità informativa. Ci si interroga sul mondo del *web* e soprattutto sulle nuove tecnologie. Queste conferiscono un carattere sempre più virtuale al mondo. Si può obiettare circa la virtualità che è una caratteristica dell'uomo, animale simbolico, ma questa diventa patologica se lo allontana decisamente dalla realtà. Come ci ha ammonito il filosofo Severino, la tecnica può essere considerata come un'espressione della natura umana tra le più belle, grandi, luminose, profonde. Essa non possiede i connotati della bruttezza e dell'idiozia soprattutto, ma maggiori sono le opportunità che offre e maggiori sono i rischi a cui espone l'uomo. Per questo l'importanza della cultura con la quale padroneggiare i mezzi la concezione dell'economia della conoscenza come un bene immateriale, che va tutelato anche dalle leggi, per capire e governare i profondi mutamenti culturali del nostro tempo, che hanno avvicinato la cultura scientifica a quella storica, attenuando il solco che separava scienza e valori, rivalutando la diversità degli individui, sono da assumere come punti cardinali per imboccare la strada giusta e risalire la china in cui il nostro Paese è precipitato per precise responsabilità politiche, non solo di questo Governo, ma di vari Governi che si sono succeduti alla guida del Paese e di vari Dicasteri all'istruzione, alla cultura e alla formazione. L'uso di Internet come mezzo culturale e didattico è importante, ma solo se si possiede una solida cultura generale che fa sì che la nostra mente sia in sinergia con il cervello, nella sua capacità di esteriorizzarsi tramite immagini e parole sotto l'influenza delle emozioni. L'uso del *web* incrementa di certo il numero dei processi e delle strutture mentali coinvolte nell'apprendimento, per cui è importante che questi strumenti si utilizzino anche nelle scuole i cognitivisti affermano proprio che l'apprendimento è migliore se si associa alle immagini. Ricorrere al materiale in rete richiede però un forte impegno e grande consapevolezza anche per quanto riguarda il corpo docente, perché il mondo del *web* non è scevro da pericoli. Le *chat* creano dei metamondi, in cui possiamo proiettare l'immagine di ciò che vorremmo essere, con il rischio però di una dipendenza e di una riduzione di contatto con la comune umanità che ci circonda: rischiamo di rimanere soli. Per non parlare poi di altri più gravi pericoli di contatto con il mondo dell'illegalità, cui la legge n. 547 del 1993 ha cercato di porre rimedio. Solo la padronanza non semplicemente tecnicistica del mezzo, ma consapevole e supportata da una robusta cultura, che non può prescindere dallo studio serio ed efficace, nell'esperienza individuale e collettiva, né dalla lettura di testi, siano essi scolastici o no, può aiutarci ad evitare questi fenomeni e a far sì che si possano costruire personalità libere, perché in grado di scegliere con le armi affilate della conoscenza. Solo la consapevolezza che questa conoscenza e la cultura sono essenziali per la crescita democratica del nostro Paese, essa sola può darci le armi pacifiche che ci mettono in grado di vincere le sfide del futuro, perché chi non è in grado è in grado di comunicare e non sa cosa comunicare oggi è tagliato fuori da questo nostro mondo, dal mondo reale. Solo investendo con convinzione sul capitale umano, sull'educazione e sull'istruzione potremo competere con le società emergenti. questo, chiediamo l'impegno al Governo a ripristinare risorse per il Centro per il libro e la lettura, per i beni e le attività culturali, per le biblioteche, non solo quelle nazionali ma anche quelle scolastiche, lasciate all'intervento delle famiglie

ad arginare la deriva culturale, la superficialità, l'effetto trainante della massificazione, che è in una controtendenza assoluta con la nostra storia culturale, fatta di ingegno individuale e di creatività personale, che non può essere massificata, ma deve essere incentivata. Chiediamo, infine, che come per tante altre spese, ad esempio quelle per le palestre, anche la spesa per i libri di testo possa trovare la disponibilità del Governo perché sia resa deducibile dalla dichiarazione dei redditi. E' un atto di grande responsabilità, perché impegna il Governo direttamente nel diritto allo studio e anche perché fa emergere l'illecito sotto il profilo della disciplina della

Grazie a tutti quelli che sono qui, alla maggioranza ed all'opposizione, a quelli che ci sono, e certamente non ringrazio quelli che non ci sono.

quali valori meritano priorità nella formazione dei nostri giovani perché la loro preparazione sia la più adatta ad affrontare le esigenze dei tempi che verranno, in modo da assicurare alla società italiana un sereno futuro. Le conclusioni della mozione sono indirizzate al Governo, in particolare al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministro per i beni e le attività culturali, nonché naturalmente al Ministro dell'economia e delle finanze, che presiede alla allocazione delle risorse. Una prima serie di raccomandazioni deriva dalla considerazione del grande processo storico in cui siamo tutti immersi, il processo di globalizzazione, caratterizzato dalla sempre più serrata competizione delle economie. L'Italia, da sempre Paese di trasformazione e quindi molto attiva nel commercio internazionale internazionale (il valore complessivo annuale delle esportazioni ammonta da tempo a più del 25 per cento del prodotto interno lordo), è profondamente coinvolta in tale processo. I nostri giovani vanno per questo adeguatamente preparati. È indispensabile prima di tutto un serio apprendimento della lingua inglese, lingua divenuta da tempo lo strumento del commercio mondiale. Ugualmente necessaria è una buona conoscenza dei mezzi di comunicazione informatici, prima di tutto Internet. Per entrambe queste esigenze la nostra scuola primaria si è organizzata da qualche anno, a partire dalla riforma Moratti. Gli studi dei nostri giovani devono inoltre diventare più seri. Passi importanti in tal senso sono stati introdotti dalle disposizioni legislative del ministro Gelmini, quali la reintroduzione della possibilità di bocciatura per cattiva condotta, la reintroduzione della valutazione di scolari e studenti con il voto in decimi, la richiesta di sufficienza in tutte le materie per l'ammissione agli esami di scuola media superiore (dall'anno scolastico 2009-2010) e modalità più severe di reclutamento dei professori universitari. Nel senso di una maggiore serietà negli studi si era mosso anche il precedente ministro Fioroni, in particolare disponendo il recupero entro agosto dei debiti formativi degli studenti. in generale, in tutte le nostre scuole va promosso, molto più che nel passato, il riconoscimento del merito. La meritocrazia, oltre a stimolare nella classe una positiva emulazione, prepara assai meglio alla competizione, che sarà la regola della vita di lavoro. Ai livelli superiori di istruzione, nei corsi di laurea specialistici e soprattutto nei dottorati di ricerca scientifico-tecnici, è necessario introdurre in modo generalizzato una specifica formazione nelle discipline economiche e gestionali, che metta in grado di svolgere analisi di mercato, formulare *business plan*, nonché accedere al credito e proteggere brevettualmente le invenzioni. Una seconda serie di raccomandazioni deriva dalla considerazione del gigantesco sviluppo ormai raggiunto dalle conoscenze scientifiche e tecniche, che sono il fondamento della società moderna, detta appunto dagli storici società tecnologica. Questo immenso patrimonio di conoscenze ha reso disponibile ai cittadini una straordinaria gamma di prodotti e servizi, ma ha anche determinato una grande complessità della società e del suo funzionamento. Ne è conseguita nella gran parte dei cittadini una sostanziale incapacità di comprendere bene come funziona la società. Ciò non avveniva nella precedente società agricola, quando più o meno tutti conoscevano i processi produttivi fondamentali. Tale diffusa ignoranza costituisce un grosso problema per il funzionamento stesso delle moderne democrazie, che tendono ad affidare direttamente ai cittadini, più che in passato, la scelta di importanti opzioni programmatiche. In altri termini, i cittadini, da un lato hanno maggiore potere di decisione, dall'altro, hanno conoscenze molto inferiori al necessario per gestire tale potere. Tale grave discrepanza si presta a pericolose strumentalizzazioni da parte di tanti: pubblicitari privi di scrupoli, guru della comunicazione esagerata ed esasperata, demagoghi, sobillatori, eccetera. In particolare, pericolosa risulta l'insinuazione delle più sconcertanti paure: la paura dell'energia nucleare, la paura dell'elettrosmog, la paura dei prodotti agricoli geneticamente modificati, la paura di catastrofici cambiamenti climatici, Queste paure sono assai facile da diffondersi per la mancanza di adeguata cultura scientifica e tecnica. Tale cultura è d'altra parte assai importante anche per la gestione ottimale della propria salute, della salute dei propri cari e per vivere tutelando adeguatamente l'ambiente. Non è facile rimediare a questa carenza di conoscenza. Sul lungo periodo occorre puntare a valorizzare nelle scuole superiori la formazione scientifica e a promuovere nella società, con opportune iniziative, anche utilizzando i mezzi di comunicazione di massa, una maggiore diffusione della cultura scientifica e tecnica. Determinante a questo riguardo è l'insegnamento più profondo delle nostre scuole, quello che sviluppa nei nostri giovani spirito critico ed autonoma capacità di valutazione, caratteristiche fondamentali della civiltà occidentale strutturatesi nei secoli con il contributo di migliaia di filosofi e giuristi nell'alveo delle grandi culture greca e romana. Una terza serie di raccomandazioni deriva dalla considerazione della grande importanza del saper leggere e del saper scrivere. Una volta si andava a scuola per imparare a leggere, scrivere e far di conto. Nonostante l'enorme facilitazione dell'accesso agli studi che si è verificata in questi decenni, l'avvento della televisione sta pericolosamente allontanando i nostri giovani dalla lettura e dalla scrittura. La lettura è un'azione assai complessa dal punto di vista cerebrale. Occorre conoscere il significato delle singole parole che si leggono e riuscire a collegarle nel cervello per riprodurre la scena che la frase vuol rappresentare, tenendo conto anche delle frasi precedenti. La corteccia cerebrale, con tutto il suo enorme patrimonio di esperienze, è impegnata a fondo nella lettura sia nell'emisfero sinistro sia nell'emisfero destro. Al contrario, la visione di una scena, in particolare la visione della televisione, è per il nostro cervello assai più agevole. In termini più banali, è molto più facile guardare la televisione che leggere un libro. Ma la televisione sviluppa poco fondamentali capacità di cui abbiamo tanto bisogno, la capacità di astrazione, di sintesi, di valutazione critica, e indebolisce la fantasia. Il susseguirsi televisivo di una scena dopo l'altra non facilita le pause di riflessione e di astrazione dalla scena, che ne consentono una sua più profonda collocazione e valutazione, e tende a determinare un atteggiamento passivo nella persona. L'allontanamento dalla lettura (e a maggior ragione dalla scrittura) prodotto sui nostri giovani dalla televisione tende purtroppo a protrarsi nella vita adulta. Il nostro cervello ha una grande plasticità, ma questa straordinaria capacità purtroppo decresce con il passare degli anni. Un solo esempio: una lingua si impara a parlare come madrelingua solo sotto i 10-12 anni. Successivamente, non si riescono più a memorizzare con la necessaria finezza le complesse sequenze muscolari che presiedono nella cavità vocale alla creazione dei suoni delle parole. Per la lettura vale un analogo discorso. Occorre imparare a leggere prima possibile. Più tardi diventa troppo difficile e faticoso. Da qui l'importanza di una scuola che non solo insegni a riconoscere le lettere dell'alfabeto, ma faccia amare la lettura. Un discorso ancora più complesso è quello dello scrivere. Scrivere richiede capacità di organizzazione ordinata non solo del pensiero della singola frase, in cui il soggetto, le sue specificazioni, il verbo (nella varietà delle articolazioni espressive), l'oggetto dell'azione, tutte queste parti della frase devono essere ciascuno al suo posto secondo le regole precise per dare significato; ma anche l'architettura delle frasi nel complesso del pensiero che si vuole esprimere deve improntarsi a coerenza, chiarezza, ordine. Anche lo scrivere va imparato presto, altrimenti non si impara più. E lo scrivere rappresenta la modalità più profonda e precisa che noi abbiamo di comunicazione e di approfondimento. Il filosofo Popper ha scritto pagine famose sul rischio che nei nostri giovani una visione quotidiana di televisione, eccessiva e sregolata (con continui episodi di violenza), possa determinare una vera e propria catastrofe formativa. Di grande importanza per i nostri giovani sono i valori etici che la civiltà occidentale, con il contributo determinante delle religioni giudaica e cristiana, ha saputo strutturare e inserire nel DNA della nostra società. Infine, va sottolineata l'esigenza, nei corsi di studio, di un'adeguata attenzione a unire alla formazione al fare, il rispetto e la promozione del bello, della qualità estetica del fare. Con queste premesse, si comprendono bene le raccomandazioni al Governo di questa mozione: il rafforzamento nelle scuole di ogni ordine e grado della massima serietà degli studi; l'adozione nella scuola secondaria superiore e nell'università di criteri meritocratici nella valutazione sia degli studenti che dei docenti; lo sviluppo e l'adozione di nuove modalità di supporto all'insegnamento, in particolare utilizzanti i programmi telematici di *e-learning* come i progetti delle LIM (Lavagne Interattive Multimediali) che, laddove sono state applicate, sono risultate di straordinaria efficacia; il sostegno, con adeguati finanziamenti, alle attività del Centro per il libro e la lettura, operante presso la Direzione generale per i beni librari, gli Istituti culturali e il diritto d'autore del Ministero dei beni e le attività culturali; l'adozione di una programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo molto più attenta di quanto non sia attualmente alle esigenze di formazione dei nostri giovani; l'intervento, con opportune iniziative e finanziamenti, al sostegno di processi di digitalizzazione del patrimonio bibliografico italiano, con particolare riferimento al programma Biblioteca digitale italiana, in modo da facilitare l'accesso a tale patrimonio in sintonia con lo sviluppo dei mezzi di comunicazione elettronici; infine, lo sviluppo nei principali musei del Paese di moderne modalità di presentazione dei tesori artistici contenuti, che ne facilitino per il pubblico giovanile l'inquadramento, la comprensione e l'apprezzamento. *(Applausi

Gruppo dell'Italia dei Valori ha presentato una mozione sulla necessità di una maggiore attenzione alla formazione culturale dei giovani e la illustro ora molto sinteticamente. Il secolo appena concluso ha profondamente mutato il concetto di cultura. Volendo definire il significato attuale del termine cultura, occorre tener presente che esso non può essere ricondotto a canoni predefiniti e immutabili. Possiamo, però, oggi distinguere tra due accezioni: la prima riguardante la possibilità di coltivare la propria conoscenza e la seconda, cosiddetta antropologica, afferente all'insieme dei costumi, delle credenze, dei valori ed ideali di un gruppo sociale o etnico. In entrambi i casi, però, il bilancio statale di questo Governo è stato poco attento al potenziamento dell'istruzione e della promozione culturale, erroneamente ritenuti non portatori di ricchezza immediata. Troppo spesso, in questo anno si sono apportati drastici tagli al settore afferente l'università, la scuola pubblica e la promozione di eventi culturali. Nel primo anno di questa legislatura, attraverso le leggi nn. 133 e 169 del 2008 così come la n. 1 del 2009, sono stati ridotti gli stanziamenti precedentemente previsti dal bilancio dello Stato. Per esempio, nel settore della scuola primaria il quarto Governo Berlusconi ha soltanto ridotto l'organico docente, mettendo a serio rischio la qualità dell'offerta formativa. Allo stesso modo, al settore universitario sono state destinate poche risorse alla realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali e non. I dati delle recenti statistiche parlano invece chiaro: proprio quando le persone sono più attive dal punto di vista lavorativo, tra i 25 e i 44 anni, solo il 16 per cento di esse fa letture professionali. I dati a disposizione consentono di smentire inoltre l'opinione diffusa che i più giovani leggano poco: bambini e ragazzi sono i maggiori lettori e il problema è la disaffezione al libro man mano che passano gli anni. È vero invece che bambini e ragazzi italiani leggono molto meno rispetto ai coetanei europei, cosa che vale anche per gli adulti. Dobbiamo anche rilevare che siamo ai livelli più bassi in Europa per la conoscenza delle lingue straniere; anche per quanto riguarda le nuove tecnologie l'Italia non è certo ai primi posti in termini di penetrazione di Internet nelle famiglie e nelle aziende e nell'alfabetizzazione informatica in genere. La formazione culturale delle generazioni più giovani riveste invece un ruolo fondamentale al fine dell'acquisizione delle informazioni, delle conoscenze e delle competenze per affrontare con capacità critica la complessità di un mondo multiculturale, dai confini sempre più vasti. La creazione di nuove biblioteche scolastiche pubbliche e l'implementazione di quelle esistenti con gli strumenti informatici più comuni ed utili, così come le iniziative volte alla maggiore divulgazione dei testi in genere, rivestono carattere di primaria importanza al fine della promozione del sapere nel nostro Paese. La promozione di un sapere pubblico, laico e bilanciato nell'analisi delle diverse esperienze storico-politiche, culturali e religiose del Paese, non può in alcun modo essere oggetto di condizionamenti di parte o di tagli indiscriminati sotto il profilo finanziario.

a promuovere una massiccia informatizzazione delle strutture che ospitano le scuole e le università pubbliche; a destinare maggiori risorse economiche al settore della scuola primaria e secondaria al fine del miglioramento e della sicurezza delle infrastrutture e dell'aumento dell'offerta formativa; a valutare un significativo aumento delle risorse economiche da destinare alle università pubbliche, al fine di migliorare l'offerta formativa oggi presente, di ampliare i campi di ricerca finalizzata allo sviluppo, di implementare le strutture da sempre drasticamente scarse da destinarsi alla fruizione dei servizi legati all'istruzione superiore. *(Applausi Signora Presidente, l'Europa, per competere a livello globale, deve potersi imporre con un'economia basata sull'innovazione, i saperi e la conoscenza. Un'economia che per essere sostenuta ha bisogno di cittadini consapevoli e attivi attraverso la valorizzazione dei diritti-doveri di cittadinanza e della pratica dell'inclusione sociale. I veloci cambiamenti che avvengono giorno dopo giorno, il passaggio dalla comunicazione testuale a quella digitale, la continua innovazione tecnologica e la globalizzazione hanno imposto la necessità di imparare ad apprendere durante tutto l'arco della vita, a confrontarsi con le diversità, con percorsi cognitivi estremamente dinamici e quasi obbligatoriamente ricorrenti. Viviamo in un'epoca nuova dove non esiste più la divisione tra una fase della vita in cui si studia e una fase in cui si lavora. Lavoro ed apprendimento, cittadinanza e dinamiche sociali, partecipazione e *governance* si fondono continuamente tra di loro, aprendo nuove grandi opportunità ma anche nuove grandi criticità. Siamo in un'epoca in cui prevale l'elemento tecnico; nell'era della seconda rivoluzione tecnologica, quella digitale, il concetto di funzionalità impone che prevalga tutto quanto sia coerente con questa visione del mondo: prevale l'inglese perché lingua tecnica efficace, prevale la comunicazione breve degli SMS e delle *e-mail*, prevalgono i manuali sui testi, le istruzioni d'uso Tutto ciò richiama il bisogno, non di opporsi a tali processi che sarebbe assolutamente impossibile, ma di sostenere nel contempo anche le forme di comunicazione: la lettura, il gusto per l'approfondimento, il confronto culturale, la valorizzazione della qualità del testo e dei contenuti ed anche, facendo una traslazione di intenti, di tutte le forme di espressione artistica. Ciò per motivi culturali, per tutelare la diversità che ha sempre un valore positivo, contrastando l'impoverimento comunicativo e l'omologazione, perché oggi conoscere più lingue è assolutamente fondamentale per l'ingresso nel mondo del lavoro, tanto più in un Paese come l'Italia in cui l'economia turistica svolge un ruolo fondamentale. Anche l'editoria risente di tale mutamento: pensiamo solo al grande cambiamento imposto dall'esplosione del *web*. Occorre sostenere la piccola e media impresa editoriale, almeno quando questa è segnata dalla qualità, da una specializzazione che non sempre la grande impresa è in grado di perseguire. Aiutiamo a confrontarsi con l'innovazione nell'editoria vera e propria, nell'utilizzo della multimedialità, nel confronto del *web*, promuovendo e sostenendo la lettura, in modo particolare tra i giovani. Scuola, formazione professionale ed approfondimento non formale nei luoghi di lavoro sono le articolazioni attraverso le quali si strutturerà il sistema del *long life learning*, un sistema che in Italia va ancora in gran parte plasmato e che, soprattutto, è ancora lontano dal rispondere alle nostre esigenze. discussione, indicando alcune linee di intervento per l'editoria, la comunicazione, il rinnovamento tecnologico ed alcune priorità, come l'invito alla lettura per i giovani e il sostegno alle famiglie, come ha sottolineato anche la collega Sbarbati, si propone di impegnare il Governo a collocare i suddetti temi al centro dell'attenzione politica. Tra le proposte, una è particolarmente concreta, ossia quella di verificare la possibilità di rendere la spesa per i libri dei testi scolastici deducibile dal reddito delle famiglie,

In particolare, mi ha molto persuaso l'obiettivo della mozione illustrata dal collega Possa, la quale rivendica due punti che vorrei richiamare, perché ci introducono ai temi più specificamente inerenti il mondo del libro, richiamati Possa ed altri colleghi si richiamano ai valori della serietà degli studi nelle scuole di ogni ordine e grado e, per non essere generici, fanno un riferimento, nel nel secondo punto, alla scuola secondaria superiore e all'università, e all'esigenza di resuscitare criteri meritocratici. Se così fosse, i confini fra libri di testo e altri libri sarebbero molto più sfumati che non nelle argomentazioni sviluppate dalla collega senatrice Sbarbati. infatti che la scuola italiana sia stata sconfitta nell'impatto con la società di massa perché ha creduto che una scuola di massa potesse abdicare ai due punti della mozione del senatore Possa; invece, è esattamente il contrario e se ne trova riscontro proprio nelle produzioni editoriali.

ad Abbagnano o a De Ruggiero. Quelli sono libri. Questa dogmatica un po' catechistica del libro di testo,

è una ferita a qualsiasi idea del libro. Se vi sono specificità dei libri di testo rispetto ad altri libri, non è la promozione della cultura il momento nel quale le dobbiamo mettere al centro della nostra attenzione. Ben venga poi ogni progetto di biblioteca digitale questo rivolgermi specificamente al sottosegretario Pizza, qual è la politica del Governo sul sistema di biblioteche? È una politica, a mio giudizio, vile e rinunciataria, in cui il cedimento al cosiddetto mondo delle autonomie e delle Regioni è fatto di un'abdicazione colpevole, 24 luglio 1977, n. 616, di Massimo Severo Giannini. Che lo Stato abbia soltanto biblioteche di conservazione del reticolo attraverso l'istituto delle sovrintendenze, è stata una politica miope e sbagliata, che ha portato poi le biblioteche di conservazione a doversi aprire al pubblico di massa delle tesi di laurea, che sono la morte civile di ogni istituto bibliotecario.

prima una scuola di qualità e poi una società che dà valore alla cultura invece che all'apparire, al solo produrre e al solo reddito? L'alfabetizzazione è uno degli strumenti che servono a combattere la povertà, povertà mentale ma anche materiale, con l'alfabetizzazione e con l'acculturarsi, con l'essere curiosi, con l'approfondimento; altro che *long life learning*, sono stati tagliati i fondi per le scuole serali, non solo per i corsi per adulti! Si è parlato di inglese potenziato in mano ad insegnanti unici, con 150 o 200 ore di aggiornamento.

prescinde completamente da un approfondimento socio-educativo, pedagogico, neuro-psichiatrico e neuro-psicopedagogico-pediatrico: ci siamo trovati di fronte ad un insegnante

Abbiamo discusso di scuola in 60 giorni, quando ci è andata bene. Il Governo ha posto delle fiducie e abbiamo parlato di risparmio, non di scuola. La scuola diventa di qualità se riteniamo di inserire in quell'ambito privilegiato tutte le sollecitazioni possibili.

altre materie ha tutti sei, che è stato svogliato, ad un bambino che semplicemente non ha dato fastidio, sia un modo per valorizzare il merito. La circolare del Ministro ha ribadito che il voto in condotta fa media. Speriamo che il dibattito di questa mattina serva anche a far correggere la circolare n. perché il mantenere ignoranti genera obbedienza e il Parlamento di un Paese democratico credo debba tenere a che la scuola sia la sede in cui si forma il cittadino, capace di intendere e di volere, di essere critico e di essere un democratico.

«impegna il Governo» aggiungere le altre «nell'ambito degli obiettivi di finanza pubblica e attraverso la riqualificazione della spesa». Al terzo paragrafo

Signora Presidente, la nostra mozione ha come obiettivo la crescita e la formazione culturale dei nostri ragazzi, futura generazione di cittadini non più solo italiani ma europei, che sempre più devono essere all'altezza della complessità del mondo che li circonda se vogliamo che l'Italia non diventi il fanalino di coda dell'Europa. I nostri ragazzi, i nostri giovani, saranno la società del futuro la loro formazione riveste un ruolo fondamentale perché possano acquisire quelle necessarie informazioni, conoscenze e competenze per affrontare, con capacità critica, la complessità di un mondo multiculturale, dai confini sempre più vasti. Se è vero, come si legge in molti studi sulle nuove generazioni, che siamo passati dalla generazione di Gutenberg a quella dei nativi digitali giovani nati e parte integrante di una società neo-tecnologica - contro ogni previsione, l'ultimo rapporto del CENSIS sulla comunicazione ha messo in evidenza il nuovo interesse dei giovani italiani per la lettura.

Quindi, se è vero che i giovani sono molto interessati e utilizzano le nuove tecnologie, è anche vero che sono in grado di passare da un mezzo di comunicazione all'altro senza fare troppo caso alla sua natura. Segno che l'utilizzo di Internet non esclude la "tecnologia" libro ed infatti, tra l'altro, il rapporto del CENSIS registra che circa il 67 per cento dei ragazzi dai 13 ai 19 anni si dichiara poco o per niente d'accordo rispetto all'affermazione che il libro di testo può essere sostituito da Internet. Il problema è stato affrontato anche dall'Associazione italiana degli editori a Roma, in occasione degli Stati generali dell'editoria 2008, dove è emerso che da qualche anno il mercato del libro segna una fase di rallentamento. Le cause sono molteplici, ma una di queste è sicuramente il costo dei libri, che spesso è molto alto, e quindi la spesa della famiglia per la cultura, da un decennio circa, è in decremento. Eppure gli esperti sostengono che è proprio il contesto familiare a favorire il contatto e il rapporto con il libro. Per questo, anche alla luce dell'attuale crisi economica, è fondamentale sostenere le famiglie per queste spese. Condividiamo, quindi, il dispositivo della mozione della collega Sbarbati: da un lato, aiuti all'editoria per investimenti in innovazione tecnologica, visto che si trova ad affrontare un mercato molto molto concorrenziale a causa della sempre maggiore egemonia della lingua inglese e di Internet e, dall'altro, un sostegno alle famiglie per l'acquisto di libri, soprattutto quelli scolastici, in particolare della scuola dell'obbligo. l'altro, che in Europa l'Italia è uno dei pochi Paesi che non fornisce gratuitamente i libri agli studenti della scuola media inferiore. Ci trova, quindi, completamente d'accordo la proposta di detassare l'acquisto dei libri scolastici per venire incontro alle esigenze delle famiglie, soprattutto di quelle più in difficoltà. E chiediamo al ministro Gelmini che, nel passaggio all'*e-book*, il libro scolastico in formato elettronico, non si dimentichi di tutte quelle famiglie e dei loro ragazzi che non si possono permettere l'acquisto di un computer e che rischiano di dover fare migliaia di pagine di fotocopie. Riteniamo fondamentale l'istituzione di biblioteche scolastiche, la promozione di nuove biblioteche pubbliche e l'aggiornamento delle esistenti, arricchendole anche di nuovi strumenti tecnologici. Non è più possibile lasciare al privato, alle famiglie, tutto il peso economico della spesa per la preparazione culturale dei nostri ragazzi. Infatti oggi può considerarsi fortunato quel bambino o ragazzo che nasce in una famiglia in cui ci sono libri, in cui i genitori sin dall'infanzia non solo hanno acquistato, ma hanno letto per lui storie e fiabe, determinando così il suo futuro di lettore e di cittadino. Ma questa opportunità deve essere data a tutti e quindi lo Stato e le istituzioni, non solo il privato, se ne devono far carico e considerare la spesa per la formazione e l'istruzione non un costo, ma un investimento per il futuro del nostro Paese. La cultura richiede investimenti, non i tagli effettuati fino ad oggi da questo Governo. E' importante che si coltivi e si promuova sempre più la cultura nel nostro Paese se si vuole tornare ad avere quell'autorevolezza culturale che, in passato, tanti ci riconoscevano e se vogliamo che l'Italia abbia dei futuri cittadini che siano il volano della nostra economia. Per queste ragioni, invito i colleghi a esprimere un voto favorevole alla mozione

Signora Presidente, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, la Lega Nord pone, da sempre, grande attenzione alla cultura del territorio, radicata nelle tradizioni popolari, attraverso la valorizzazione delle lingue locali, di usi e costumi, dei repertori teatrali, musicali e letterari del posto. Non a caso ci battiamo contro uno Stato centralista che per forza di cose passa come un rullo compressore su un territorio come quello del nostro Paese, che custodisce oltre il 60 per cento di tutte le opere d'arte mondiali. Un vero affronto alla cultura. Con il federalismo siamo tesi al recupero del vissuto identitario dei popoli da cui discendiamo. Un patrimonio da non disperdere, in tempi di globalizzazione e massificazione culturale estrema, che tende all'annullamento delle identità, quando invece è proprio un'identità forte a consentire la sopravvivenza culturale, oltre che economica. I progetti di legge presentati dalla Lega Nord hanno questo obiettivo. La cultura umanistica e la letteratura locale sono puntualmente oggetto di promozione, memorizzazione e divulgazione da parte delle nostre amministrazioni. Azioni simili vengono svolte per la musica e le arti figurative, favorendo ad esempio concerti e mostre ispirate ad autori e artisti nati e cresciuti nelle nostre terre. Riteniamo che soprattutto la televisione, che entra costantemente e, in alcuni casi, prepotentemente nelle nostre case, debba dedicare più attenzione alla valorizzazione del vissuto locale e della sua cultura. Ci rivolgiamo in particolare al servizio pubblico. Assistiamo invece a un progressivo appiattimento della TV di Stato sui modelli proposti dalle televisioni commerciali. L'obiettivo è l'*audience* a tutti i costi per soddisfare gli *sponsor* su programmi che producono «imbarbarimento culturale» nelle menti più facilmente manipolabili: quelle dei nostri giovani e delle persone che non dispongono di un adeguato bagaglio culturale, senza quindi gli anticorpi necessari per contrastare certi messaggi. Chiediamo l'impegno del Governo per favorire una programmazione televisiva sensibile e attenta allo sviluppo mentale e culturale delle nuove generazioni. Chiediamo inoltre l'impegno a favorire l'adozione di criteri omogenei nella valutazione di studenti e docenti nella scuola, dopo aver ottenuto l'attribuzione di almeno una parte dei finanziamenti alle università sulla base di criteri meritocratici onde porre fine alle sperequazioni nella destinazione delle risorse tra università del Nord e quelle del Sud del Paese. Ricordo anche che sono in arrivo fondi per borse di studio a favore degli studenti più meritevoli e per l'inserimento di nuovi ricercatori al fine di consentire un ricambio generazionale dei docenti, nonché per la costruzione di alloggi e residenze universitarie. A tale proposito, auspichiamo controlli ferrei ed inflessibili sulla qualità di queste costruzioni, al fine di scongiurare altre tragedie come quelle della Casa dello studente dell'Aquila; in quegli alloggi è custodito il nostro futuro. In conclusione, confermo il voto della Lega Nord alla mozione sulla cultura n. 129, a cui il presidente Bricolo, la collega Aderenti ed io, insieme ai colleghi della maggioranza abbiamo apposto la firma, condividendone gli intenti.

disponibili a cogliere il significato e il senso importantissimo sotto il profilo politico e culturale del dibattito che si sta svolgendo e del contenuto delle mozioni che sono state presentate, in particolare, della mozione che ho presentato a nome del Partito Democratico. Il fatto che il Governo accolga questa mozione nei suoi contenuti culturali, politici e anche d'impegno amministrativo e politico, ci fa piacere e spero sia l'inizio di una controtendenza nei confronti del sistema culturale del Paese, del sistema Paese *tout court*, nella sua connotazione e nel suo profilo di dignità culturale, che in questo momento non è troppo evidente. I rapporti internazionali che ci collocano all'ultimo posto, anche in Europa, come numero dei laureati, penultimi soltanto rispetto alla Romania, non ci possono confortare. Così come non ci confortano i dati sulla lettura. Si diceva poco fa che i bambini leggono più dei adulti, che i nostri bambini leggono forse non meno che gli altri bambini europei, ma in realtà più si cresce più la disaffezione verso il libro aumenta perché si privilegiano altri tipi di linguaggio, che sono importanti e significativi nel mondo interattivo della comunicazione e della socialità. Ciò non toglie che quello che abbiamo voluto evidenziare è che un aiuto alla cultura passa attraverso l'incentivazione alla diffusione del libro e della lettura consapevole, della lettura consapevole, che significa tutto ciò che è stato detto: dal significato delle parole alla loro etimologia, alla loro comprensione più profonda e interattiva con altre parole e linguaggi, alla capacità di comunicare e di farne tessuto fondante della propria personalità. Certamente questo può avvenire soltanto se c'è un impegno serio sotto il profilo amministrativo e politico da parte del Governo e dei Ministeri di competenza.

siamo reciprocamente riconosciuti, a nome anche dei rispettivi Gruppi, in questa battaglia che non è né di destra né di sinistra. La battaglia per la crescita culturale di un popolo e di un Paese, per la sua dignità nel contesto internazionale in cui deve inserirsi con le armi vere della conoscenza, quelle che possono portare la pace, lo sviluppo, la capacità di risollevarsi sotto il profilo della ricerca scientifica, tecnologica ed essere all'altezza dei tempi

le poste in gioco per la cultura e la formazione non subiscano i tagli che, invece, sono stati accettati in maniera pedissequa come se fossero

è assolutamente improponibile. Manifesto, quindi, apprezzamento per la decisione del Governo, che spero costituisca una svolta anche soprattutto per questo settore,

su cui venivano allocate le risorse è stato cancellato. Mi fa piacere che il Governo accolga quello che il presidente Possa ed io abbiamo sottolineato e che questo centro possa essere adeguatamente finanziato perché in quella sede si potranno fare le politiche serie che,

gli voglio ricordare che per la maggior parte delle famiglie italiane i soli libri presenti in casa sono i libri di testo scolastici.

e rivisto: questo è il libro di testo. Coniugare la storia solo al presente e non scavare negli anni passati, nel '68, per esempio, e nel deserto che quel movimento ha lasciato dietro di sé è un vecchio metodo, proprio di una vecchia politica. L'analisi di un evento storico quale il '68, se esaminata alla luce di una coscienza critica, costituisce la chiave di lettura per capire ed intervenire nel nostro tempo e ciò vale per i ventenni, per i trentenni etichettati, oggi, come generazione invisibile, domestica, contrassegnata dal disincanto politico, dal ripiegamento nel privato, senza riferimenti identitari, culturali e sociali,

Non mancano, anzi, coloro che ritengono che sia un modello da riconsiderare, con gli opportuni emendamenti ed adeguamenti, per estrarne nuove ispirazioni e valori. Invece non è così: non ci si accorge, infatti, che per recuperare e riscattare importanti valori sociali, formare le nuove generazioni, ridare loro fiducia nei grandi valori di libertà e democrazia, occorre dare esempi di testimonianza, spendersi nei propri impegni, senza ripetere gli errori massimalistici, utopistici, a volte terroristici del '68. In questo senso, ritengo che il settore della cultura debba divenire, oltre che strumento per la produzione individuale e collettiva, fattore importantissimo di coesione sociale, nonché operatore attivo dei meccanismi di sviluppo economico. Va detto e ricordato che bisogna pensare la cultura non più in termini settoriali e secondo uno schema totalizzante di conoscenze ed erudizione, ma piuttosto come sistema complesso ed interrelato, in cui diverse tipologie di acquisizione del sapere e diverse modalità di competenze concorrono in un'azione di promozione reciproca. Una scuola che voglia fare cultura deve riconsiderare, come sta facendo il ministro Gelmini, il concetto di meritocrazia e di valutazione, il quale non può essere punitivo, ma neppure esorcizzato o abolito. Esso serve piuttosto a misurare il rapporto costi‑benefici sia nella scuola che nelle università ed è un buon veicolo per innalzare la qualità dei contenuti culturali, la reale consapevolezza delle proprie conoscenza intese - esse sì come approfondimento e capacità critiche, che non possono prescindere da un percorso che comprenda la lettura di testi che aiutino il mondo giovanile a conoscere, a convivere e a dialogare con culture e civiltà diverse. L'ottica in cui si è sempre mossa la sinistra è stata quella dei documenti, dei progetti ingenti, massicci, voluminosi, ma puramente astratti.

di un provvedimento che si avvale della tecnologia informatica per abbattere i costi dei libri di testo per scuole e famiglie: vale a dire dell'adozione dei libri di testo con cadenza quinquennale ed individuazione, da parte degli organi scolastici competenti, dei siti nella rete Internet che li renda in tutto o in parte disponibili. Ricordo a tutti quando il presidente Berlusconi per la prima volta lanciò le tre

proprio per potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi limitati di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie. È anche in questo modo che intendiamo arginare la congettura e il tanto conclamato teorema della deriva culturale, sempre agitato dalla sinistra quando è all'opposizione e così arrogantemente ignorato invece quando è maggioranza. Concludo questo mio intervento

Signor Presidente, colleghi senatori, signor Vice Ministro, vorrei anzitutto esprimere il mio apprezzamento per la condivisione

La Carta europea dei diritti del malato è un documento tradotto in 22 lingue in cui vengono espressi i diritti irrinunciabili del paziente che ogni Paese dell'Unione europea dovrebbe tutelare e garantire. È il risultato di un lavoro di decine di associazioni di assistiti e consumatori europei che hanno siglato la nascita della Carta a Bruxelles nel novembre del 2002, in un incontro che ha cercato di tracciare l'identikit del paziente del futuro. Le istituzioni europee hanno accolto con estremo favore la promozione di questa Carta: dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea al Parlamento europeo, con due risoluzioni del 2007, al Comitato economico e sociale europeo, che ha espresso parere favorevole. L'esigenza di mettere per iscritto questi princìpi nasce dalla constatazione che i sistemi sanitari in Europa sono un po' lo specchio del federalismo sanitario italiano: a seconda di dove si risiede si ha accesso o meno a certe prestazioni, con tempi e livelli di qualità molto diversi. Il testo ribadisce quanto la maggior parte delle legislazioni nazionali prevedono, ma spesso dimenticano o hanno lasciato in sospeso. L'elenco contiene vecchi e nuovi diritti: dal consenso informato all'equo accesso alle cure, a quelli più innovativi come quello di evitare sofferenze e dolore non necessari. Esigenza, questa, apparentemente scontata ma che, in Italia, fa fatica ad entrare, visti i ritardi che si sono accumulati sul fronte per esempio delle cure palliative. Ritardi che noi speriamo siano presto sanati da un *iter* veloce della legge sulle cure palliative in discussione alla Camera dei deputati. I diritti sanciti dalla Carta europea dei diritti del malato sono 14: diritto a cure preventive, all'accesso, all'informazione, al consenso, alla libera scelta, alla *privacy* e alla confidenzialità, al rispetto dei tempi dei pazienti, al rispetto degli standard di qualità, alla sicurezza, alla innovazione, ad evitare sofferenze e dolori non necessari, a trattamenti personalizzati, al reclamo e al risarcimento. Con una frase si può riassumerne lo spirito: il miglior paziente è un paziente informato che, come tale, ha diritto a ricevere tutte le informazioni e la documentazione sanitaria di cui necessita, nonché ad entrare in possesso degli atti necessari a certificare in modo completo la sua condizione di salute. Ha diritto a vedere rispettato il suo tempo al pari di quello della burocrazia e degli operatori sanitari. E chiunque si trovi in una situazione di rischio per la sua salute ha diritto ad ottenere tutte le prestazioni necessarie alla sua condizione e ha altresì diritto a non subire ulteriori danni causati dal cattivo funzionamento delle strutture e dei servizi. Il Servizio sanitario ha il dovere di proteggere in maniera particolare ogni essere umano che, a causa del suo stato di salute, si trova in una condizione momentanea o permanente di debolezza, non facendogli mancare per nessun motivo e in alcun momento l'assistenza di cui ha bisogno. Il Servizio sanitario deve garantire la certezza del trattamento nel tempo e nello spazio, perché il paziente non deve essere vittima degli effetti di conflitti professionali e organizzativi, di cambiamenti repentini delle norme, della discrezionalità nella

farlo guarire e migliorare comunque sia il suo stato di salute, vedendo anche riconosciuta la sua specificità derivante dall'età, dal sesso, dalla nazionalità, dalla condizione di salute, dalla cultura e dalla religione, e a ricevere di conseguenza trattamenti differenziati a seconda delle diverse esigenze. La Carta non dimentica il ruolo della famiglia che si trova ad assistere un suo componente e per questo ha diritto di ricevere il sostegno materiale necessario. Molto importante, infine, soprattutto alla luce delle ultime discussioni parlamentari, è ricordare che la Carta garantisce il diritto del cittadino, sulla base delle informazioni in suo possesso e fatte salve le prerogative dei medici, a mantenere una propria sfera di decisionalità e di responsabilità in merito alla propria salute e alla propria vita e, anche se condannato dalla sua malattia, ha diritto a trascorrere l'ultimo periodo della vita conservando la propria dignità, soffrendo il meno possibile e ricevendo attenzione e assistenza. Colleghi senatori, l'impegno che chiediamo al Governo è quello di recepire questi diritti essenziali, ma gli chiediamo anche di svolgere un ruolo internazionale di *leadership* e di farsi promotore, nelle sedi comunitarie e in tutti i paesi dell'Unione europea, di iniziative destinate a garantire una comune ed uniforme adozione dei princìpi della Carta europea dei diritti del malato.

ad opera di organizzazioni civiche dei Paesi membri, sono sicuramente diritti fondamentali e devono essere riconosciuti e rispettati in ogni Paese; essi sono correlati con doveri e responsabilità che sia i cittadini che gli altri attori della sanità devono assumere. Chiedo quindi al Governo italiano di adottare iniziative per darsi uno strumento guida, individuando i principali diritti e doveri del paziente

Grazie a tutti In Europa, analogamente a quanto succede in Italia, i sistemi sanitari nazionali sono organizzati dagli Stati membri sulla base delle esigenze dei rispettivi cittadini; sempre più spesso però, per ragioni di vicinanza, di specializzazione nelle cure o di maggiore disponibilità delle strutture, l'assistenza viene ad Paese diverso da quello di appartenenza. È quindi importante organizzare un'assistenza sanitaria transfrontaliera più efficiente, un modello capace di promuovere innovazione e garantire a tutti l'impiego delle risorse e la qualità delle cure offerte, ed è assolutamente doveroso che anche l'Italia si adegui immediatamente.

ad oggi l'attività del Ministero è sicuramente finalizzata, anche con l'ausilio di enti di primaria rilevanza del Servizio sanitario nazionale, quali l'AGENAS (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), a garantire

A titolo di esempio, comunico che è stato avviato dal Ministero un imponente lavoro di coinvolgimento dei cosiddetti *stakeholder* tramite il gruppo di lavoro per la sicurezza dei pazienti, che ha articolato i lavori anche in un sottogruppo, dedicato proprio al coinvolgimento delle associazioni di tutela dei cittadini, e tessendo una rete di contatti, anche sopranazionali, diretti ad assicurare l'umanizzazione dei servizi grazie alla partecipazione delle associazioni nell'organizzazione e nella valutazione delle prestazioni assistenziali. In tale ambito è stata predisposta una serie di opuscoli (7 per la precisione) per un'assistenza sanitaria più sicura; essi sono rivolti a coloro che, a vario titolo, sono impegnati nella promozione della sicurezza dei pazienti.

al Nord, di fatto, i cittadini sono penalizzati, perché, a fronte di questa continua migrazione, continuano ad allungarsi le liste di attesa degli ospedali. Credo che anche la soluzione a questo problema possa passare attraverso l'applicazione completa del federalismo fiscale, quando finalmente tutte le Regioni saranno responsabilizzate e, probabilmente, queste disparità di trattamento verranno meno. Questo è il nostro auspicio e il motivo per cui

Non so se il voto di oggi sia un voto da considerare memorabile nella storia di quest'Aula. Probabilmente la mozione, come tante altre, rimarrà negli archivi e non se ne farà nulla,

negli ospedali, alla mercé anche della burocrazia medica. Annuncio il voto favorevole e ringrazio la senatrice Bianchi e il Governo;

ancora una volta intervengo per segnalare una questione molto grave e dai risvolti ormai drammatici. Dai giornali di oggi apprendiamo che i sindacati italiani, tedeschi e spagnoli,

Termini Imerese, come è stato detto da un collega in apertura di seduta, e tagliando brutalmente forza lavoro in Campania. Per ora è solo l'ultima puntata di una brutta storia per l'industria italiana e per il nostro Mezzogiorno, della quale ci stiamo occupando da quasi un anno, portando all'attenzione del Parlamento la situazione. Ci sono cinquemila lavoratori a rischio che sono in cassa integrazione al minimo e non hanno alcuna certezza su quale sarà il loro futuro e quello delle loro famiglie. Di fronte alle giuste richieste dei sindacati, alla mobilitazione di un'intera comunità regionale a favore dello stabilimento FIAT di Pomigliano d'Arco e alla forte presa di posizione della Chiesa il Vescovo ha scritto al Governo e il Papa ha ricordato questo dramma nel suo Angelus - non c'è stata alcuna risposta da parte della certamente rafforzata dalle sue nuove alleanze economiche internazionali sul piano industriale e nella sua missione strategica, né dal Governo è stata data alcuna risposta alla richiesta di una convocazione urgente di un tavolo istituzioni-sindacati. Il Presidente del Consiglio, in una alle sue ricorrenti visite in Campania, parlo di quelle istituzionali, ha incontrato gli operai e li ha rassicurati dicendo che se ne occuperà presto. Sono trascorre tante e tante settimane e l'agenda del Governo ha dovuto occuparsi di altre priorità. Quand'è il turno di Pomigliano d'Arco? Quando serietà e concretezza prenderanno il sopravvento su questa vicenda? Se il progetto di cui si è parlato in Germania fosse vero, un ulteriore grave tradimento delle ragioni del lavoro e del Sud si perpetrerebbe. Sabato, a Torino, accompagnati dalle istituzioni locali, lavoratori e sindacati faranno sentire ancora la loro voce. Noi siamo al loro fianco. Diamo piena adesione alla manifestazione ed esprimiamo totale solidarietà per la vertenza FIAT a Pomigliano. Le chiedo, ancora una volta, Presidente,

Presidente, desidero comunicare a lei e all'Assemblea la nostra apprensione e il nostro sgomento per ciò che sta accadendo in queste ore in Birmania; lo faccio anche a nome dell'Intergruppo parlamentare «Amici della Birmania», al quale hanno aderito parlamentari di tutti i Gruppi politici. Questa mattina lo stesso intervento è stato svolto alla Camera dei deputati dalla collega Margherita Boniver.

La comunità internazionale ha condannato unanimemente la mancanza del rispetto dei diritti umani, della libertà e l'assenza della democrazia in Birmania. Siamo vicini al popolo della Birmania e lo siamo stati in modo particolare quando è arrivato il ciclone Nargis.

pensiamo che debbano farlo anche il nostro Paese - e sappiamo dei contatti che sono in atto anche in questo momento - e l'Unione europea. Occorre assicurare l'avvio di una vera transizione verso la democrazia, iniziando dalla liberazione immediata di Aung San Suu Kyi

Grazie a tutti affinché ci sia un movimento politico internazionale volto a far partire davvero in Birmania una fase nuova. Ricordo anche che in molte città italiane, governate da segno politico diverso, si è provveduto a dare la cittadinanza onoraria ad Aung San Suu Kyi e ad altri prigionieri politici della Birmania. È in nome di questa società civile italiana, oltre che della nostra concezione della democrazia e dei diritti umani universali, che oggi chiediamo che il Senato si faccia interprete presso il Governo dell'assoluta necessità di fare sentire la voce dell'Italia. In quest'Aula, il diritto, la giustizia, la fortezza, la concordia. Questa è un'Aula in cui i diritti umani universali hanno cittadinanza. Noi vogliamo affermare che tale cittadinanza appartiene a tutti i popoli ed anche a quello della Birmania, che deve essere messo nelle condizioni di vivere